una volta conclusa la seduta pomeridiana di ieri ho riunito la Giunta per il Regolamento per ascoltarne il parere in merito al denunciato contrasto tra 1'articolo 6 e l'articolo 29 del provvedimento al nostro esame. La Giunta ha convenuto che, sulla base di un esame complessivo del Regolamento, non emergono in capo alla Presidenza poteri idonei a risolvere la questione prospettata, non potendo la Presidenza stessa, nel caso di specie, pronunziare dichiarazioni di stralcio, inammissibilità o preclusione. La norma di chiusura alla quale è possibile ricorrere nella fattispecie è soltanto quella dell'articolo 103 sulle modificazioni di coordinamento, da richiedersi prima della votazione finale e da assumersi con apposita deliberazione dell'Assemblea. Il parere della Giunta è stato adottato a maggioranza.

la lettura del Resoconto stenografico e sommario chiarisce che ieri pomeriggio la Presidenza del Senato, invocando più volte specifici precedenti e dando interpretazione del comma 1 dell'articolo 118 che a nostro avviso può configurare anche una lesione delle prerogative della Presidenza di turno, ha annullato, dopo la sospensione della seduta, non solo l'ultima, bensì una quindicina di votazioni di emendamenti riguardanti commi diversi del provvedimento in esame, per i quali la Presidenza di turno, ai sensi dell'articolo 111 del Regolamento, aveva proclamato risultati differenziati, dandone alcuni per approvati ed altri per respinti, come tutte le registrazioni video dimostrano ed il resoconto sancisce in modo inequivocabile. di ieri, invece, la Presidenza di turno, interpretando lo stesso articolo 118 del Regolamento, non ha consentito la rinnovazione di votazioni dalle quali era emerso che un Ministro della Repubblica aveva votato per conto di un altro Ministro senatore. In quel caso, la Presidenza successiva non ha inteso smentire la Presidenza di turno. La richiesta pertanto è la seguente, Primo: che la Presidenza comunichi all'Assemblea gli estremi dei precedenti in cui una Presidenza diversa dalla Presidenza di turno abbia annullato non solo l'ultima votazione prima prima della sospensione della seduta, bensì oltre 10 votazioni afferenti emendamenti diversi e commi diversi di un disegno di legge aventi esito differenziato (reiezione o inammissibilità in una decina di casi e approvazione in altri quattro casi). casi). Il precedente deve essere specificato secondo questo criterio. Secondo: che l'elenco, il repertorio, il massimario o la serie, come vogliamo chiamarlo, dei precedenti, sia una volta per tutte messo a disposizione dell'Assemblea o comunque di tutti i Capigruppo, al fine di evitare che la sola Presidenza di turno possa discrezionalmente selezionarli e invocarli, senza possibilità per l'Assemblea di controllare l'esatta rispondenza del presunto precedente al caso in specie o anche la presenza di precedenti di segno opposto o diverso. Terzo: che sia chiarito in base a quali norme regolamentari si possa assumere, invocando precedenti prassi, una data decisione - attenzione! - e subito dopo affermare che essa non costituisce precedente. Quarto: che la Presidenza del Senato convochi la Giunta per il Regolamento per disciplinare le forme di accesso di tutti i senatori, o almeno dei Gruppi, al massimario dei precedenti, nonché per chiarire gli spazi di tutela delle Presidenze di turno rispetto alla Presidenza del Senato o ai turni successivi di Presidenza. In particolare, la Giunta dovrebbe ancorare a criteri precisi l'interpretazione - cui deve attenersi ciascuna Presidenza di turno sulla questione dei cosiddetti pianisti, e quindi anche sull'articolo 118 del Regolamento in relazione alla questione dell'immediatezza della rinnovazione del voto irregolare. Su tali aspetti ci sono state, ci sono state, come è noto, non solo pronunce della Corte costituzionale, ma anche deliberazioni del Consiglio di Presidenza del Senato, che è opportuno chiarire per salvaguardare la certezza delle deliberazioni dell'Assemblea che la giornata di ieri ha posto in serio dubbio, potendo la situazione che si è verificata giungere perfino ad alterare il corretto processo di formazione delle leggi, in base al quale se un testo all'esame di un ramo del Parlamento viene modificato esso deve passare all'altro ramo.

Gli Uffici, in ordine ai precedenti, le forniranno puntuali riferimenti. Le posso significare che per quanto mi riguarda, per la mia esperienza, io stesso - l'ho detto ieri e lo ribadisco ho fatto ripetere un paio di votazioni elettroniche, proprio perché non ero convinto e, quindi, ne sono testimone. Ma gli Uffici le daranno tempestiva conferma di questi precedenti, atteso comunque il fatto che nella seduta di ieri

se abbiamo l'articolo 8 del Regolamento che conferisce ad un Presidente di Assemblea un potere sull'ordine delle votazioni,

cui noi votiamo la prima norma non si può poi mettere in votazione una seconda norma, perché questo non sta né in cielo né in terra. Significa che ammettiamo che il Parlamento, nella stessa legge, possa volere e disvolere; accettiamo che il Parlamento sia schizofrenico. È una cosa mai vista in questi termini. Un conto è se c'è una contraddizione che si rileva alla fine: alla fine, ci si accorge che, non volendo, ci sono cose contraddittorie (e questo è il coordinamento formale); ma se lo sappiamo prima che ci sono due cose opposte, si rimedia prima. Altrimenti il lavoro parlamentare diventa una farsa in cui è possibile sostenere tutto e il contrario di tutto, nello stesso momento, da parte delle stesse persone. Quindi, l'idea che interveniamo sul coordinamento formale è una specie di contentino che viene dato dalla maggioranza, che poi voterà anche contro il coordinamento formale perché altrimenti il testo dovrebbe andare alla Camera. Per sopprimere il comma 11, per fare un emendamento che toglie il comma 11 da una legge, per paura dei deputati della maggioranza o di dissensi politici, o per il fatto che vogliono andare in vacanza, la maggioranza e il Governo ci fanno approvare una cosa del tutto schizofrenica. Tralascio poi le altre schizofrenie di ieri, come aver dichiarato in pubblico che si possa fare un decreto correttivo su un testo ancora non entrato in vigore. Anche questo resterà agli annali non a onore della storia del Senato. Qui siamo veramente ad una cosa totalmente insensata. Voi vi assumete una responsabilità gravissima. Mi riferisco anche all'argomento usato ieri dal presidente Quagliariello per cui, siccome c'è il rapporto fiduciario, il Governo può correggere le cose che il Parlamento non è in grado di correggere. Questo è vero se il Parlamento commette un errore e non se ne accorge, e allora si ricorre alla decretazione d'urgenza per rimediare. Ma se si sa già prima, equivale a dire: io non mi sono preparato, sono in rapporto di fiducia con il mio compagno di classe, copio il compito da lui perché abbiamo un rapporto fiduciario. Guardate che stiamo sostenendo delle cose assurde. Io mi limiterei alla logica, non al diritto, per rifiutare questa interpretazione.

non per fatto personale, ovviamente, ma per riportare un po' di chiarezza in questa materia dove ci sono degli aspetti formali e degli aspetti politici. Gli aspetti formali:

quella dell'articolo 6 e quella dell'articolo 29 - non sono tali da implicare una contraddizione logica. Io sfido chiunque a dimostrare che la volontà del legislatore non sia chiara. A questo punto, si pone un problema che riguarda il bicameralismo. Io lo dico con molta chiarezza: quel testo doveva essere corretto in sede di coordinamento dalla Camera dei deputati e ritengo estremamente grave che ciò non sia stato fatto. In questo modo, infatti, si crea un altro precedente, in virtù del quale una Camera può garantirsi, evitando un coordinamento, una lettura supplementare, il fatto che il testo gli torni, se si fissasse - come vorrebbe il collega Ceccanti - l'obbligo dell'altra Camera di supplire ad un qualcosa che era doveroso fare prima. Perché non c'è una contraddizione logica all'interno di quel testo: c'è una contraddizione formale che in sede di coordinamento si poteva risolvere. A questo punto, all'interno di un sistema bicamerale che è anche sistema parlamentare, nel quale la maggioranza e il Parlamento comunicano con il Governo, ci sono tre possibilità di intervenire su questo *vulnus*: la prima è quella di cambiare il testo; la seconda è quella di agire in sede di coordinamento; e, infine, la terza è quella di prendere atto di una volontà dell'Esecutivo di intervenire successivamente. La scelta a questo punto è una scelta politica, che evidentemente ci si assume in piena responsabilità. All'interno di questa scelta politica entrano in gioco tanti altri fattori che la maggioranza e l'opposizione hanno il diritto e il dovere di considerare,

Se la maggioranza sceglierà di non fare il coordinamento, ma di agire attraverso un impegno assunto dall'Esecutivo - ripeto che ciò è assolutamente ordinario in un sistema nel quale il potere esecutivo e il potere legislativo comunicano e non sono separati: è per questo che quando il Governo interviene in Aula si apre un dibattito che nessuno può interrompere - lo farà a volto scoperto, senza nascondersi dietro un dito e assumendosi fino in fondo la propria responsabilità politica, che in questo caso sarà quella di fare approvare una legge nella quale la volontà del legislatore non è in dubbio. *(Applausi

Non c'è nessuna contraddizione formale nel testo: la contraddizione è di merito, esplicita e netta, e tanto lo è

e che probabilmente non sarebbe in grado di ricevere quell'emendamento per inammissibilità, oppure addirittura ad un decreto-legge che sarebbe emanato dal Governo per sanare questa situazione.

può chiedere il voto di fiducia su un testo, certamente può presentare emendamenti, ma non può entrare nel recinto della regolarità del procedimento legislativo. Quando ciò accade è una spoliazione indebita. *(Applausi dal *PD)*. Tanto più se l'intervento del Governo viene annunciato mentre il procedimento legislativo è in corso di svolgimento e prima ancora che il Senato sia chiamato a deliberare sul punto.

In sede di coordinamento formale, la Camera non ha ritenuto di intervenire. Abbiamo quindi già una prima pronuncia di merito e una prima pronuncia sotto il profilo del coordinamento formale.

non va abrogato, e quindi sarà respinto il nostro emendamento. E non ci vuole molto ardimento a scommettere sul fatto che, in sede di coordinamento formale, la proposta di eliminazione di quella norma verrà respinta. Quindi, Camera e Senato si pronunceranno complessivamente due volte nel merito e due volte in sede di coordinamento formale, poi arriverà il Governo e presenterà un emendamento al decreto milleproroghe. Non so proprio di cosa stiamo parlando! È un mostro che stiamo coltivando, lo stiamo facendo crescere e coccolando, invece saremmo assolutamente in tempo per evitare che tutto questo si produca.

ha segnalato a noi senatori quali siano i limiti afferenti la possibilità che lei ha di intervenire nel corso dei lavori

- d'accordo, a maggioranza

Il problema politico sorgerebbe, come giustamente è stato detto, qualora, indicataci una strada, poi non la coltivassimo. Diventerebbe una beffa: siamo tutti convinti di una certa cosa, sappiamo con quale strumento possiamo farla e poi decidiamo di non farla. Questo sarebbe un po' prenderci in giro.

farsi interprete politico della soluzione. Il momento in cui lei ritorna in campo con la sua autorevolezza è proprio quello descritto all'articolo 103 Quindi, dal punto di vista regolamentare sono convinto del rigore e dell'esattezza della decisione assunta,

Lei giustamente ha dovuto convocare la Giunta per il Regolamento per capire il modo di procedere, senza voler fare strappi in un momento in cui il clima già non era dei migliori. Giustamente su queste norme, su cui - diciamolo - abbiamo verificato una certa incongruenza, lei si è dichiarato sostanzialmente senza mezzi propri per poter intervenire. Infatti lei, Presidente, non poteva dichiarare l'inammissibilità di queste due norme, non trattandosi di disegno di legge collegato o di comunitaria; non poteva dichiararne la preclusione, stante il fatto che non erano né emendamenti né ordini del giorno; men che meno il Presidente dell'Aula avrebbe potuto dichiararne lo stralcio, in quanto erano norme di un provvedimento arrivato in questa forma nell'Aula del Senato. Cosa deve fare il Presidente del Senato? Probabilmente rivolgersi prima alla Giunta per il Regolamento per capire la strada, poi ai Capigruppo, perché la questione diventa prettamente politica. L'unica via d'uscita, che mi pare che anche senatore Quagliariello abbia indicato e che spetta a tutti i membri di quest'Aula, è invocare il coordinamento *ex* articolo 103, che ogni senatore, senza questioni di numeri e di *quorum*, può chiedere al Presidente evidenziando, come abbiamo chiaramente percepito, l'incongruità delle due norme dell'articolo 6 e dell'articolo 29 e l'Aula si esprime sul coordinamento tecnico. Il problema si sposta tutto in sede politica, perché poi ci saranno diverse strade: l'Aula, per recepire,

approvare questo testo sapendolo imperfetto sotto il profilo normativo, considerando che anche norme incostituzionali possono essere emanate da un'Aula, salvo poi trovare l'approvazione o la cassazione in sede di giudizio di costituzionalità. Ma - e passate il paradosso - se quest'Aula può emanare norme incostituzionali, cioè norme che contrastano con una norma di rango costituzionale, figuratevi se non può emanare una norma che al limite contrasta con una norma ordinaria di pari rango. È una questione prettamente politica. Ai colleghi dell'opposizione, però, vorremmo dire che il momento del dibattito non può essere adesso sulla questione procedurale aperta dal Presidente, ma sarà dopo, prima del voto finale, caro costituzionalista Ceccanti, quando anche lei potrà alzarsi e chiedere che venga proposta, proposta, in sede di coordinamento, la revisione del testo. Fino a quel momento, il Presidente ha agito perfettamente e correttamente secondo il Regolamento.

della riunione della Giunta per il Regolamento, con l'esito non unanime del parere della stessa, che ha assistito poi la decisione che lei ha proposto all'Assemblea. Voglio puntualizzare che nell'avere espresso il mio parere favorevole all'applicazione dell'articolo 103 come strumento per dirimere questa vicenda così anomala,

arbitrale, ma mi sono anche affidato alla sensibilità e alla correttezza da lei manifestate nella gestione di un passaggio parlamentare particolarmente convulso e di difficile soluzione.

Presidente, l'esito di questa vicenda non sarà secondario nel determinare il mio voto sulla legge, perché voglio comprendere

flessibilità, ma correttamente, abbiamo enucleato la volontà dell'Aula e non fatto prevalere le condizioni accidentali che si erano determinate. Nella stessa logica, la piena consapevolezza di un

nel ribadire il mio affidamento alla sua responsabilità nella convinzione che lei non poteva precludere questa norma ma utilizzare l'articolo 103, chiedo alla maggioranza di ragionare bene

8.3 torniamo per forza su un tema cruciale. Credo che lei, come me, abbia sentito che alla nostra critica che non si può fare una riforma vera senza che ci sia un minimo di investimento

So capire, soprattutto, che questa legge si innesta su un percorso che ha visto già molto decurtate le sostanze a favore della ricerca, dell'università e della scuola in Italia, per cui ciò che è stato introdotto non è aggiunto: mancano ancora fondi, e se questa è una legge ordinamentale, mi chiedo come mai non siamo riusciti ad ottenere ciò che il Ministro aveva annunciato in una delle sue presenze in Commissione, cioè di fare una legge di prima norma. Sarebbe stato bellissimo, perché ogni giovane, ogni famiglia, noi stessi avremmo letto dalla prima all'ultima riga il testo di una legge che doveva allargarci il cuore,

la Camera fortunatamente li ha ripristinati, cosicché un Gruppo di recente formazione ha potuto votare la legge e comunque, dopo che ha ottenuto tanto, senatore Valditara, poteva anche chiedere di stabilire almeno un'idea di come finanziare il provvedimento. Lei ricorda spesso il mio disegno di legge: ebbene, in esso c'era un fondo istituito con la capacità, anno per anno, di integrarsi, dando garanzie alle università, la cui autonomia significava anche sapere che preventivi fare e che consuntivi approvare. A furia di non prevedere nuovi oneri, nessun onere, non so come questa legge, che pure sarebbe stata utile al Paese, potrà diventare effettivamente attuabile. Per questo motivo, un emendamento così sobrio, signor Presidente, riguarda interamente lo spirito

*(PD)*. Signor Presidente, l'articolo 8 riguarda la revisione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari e quindi approfitto di questa dichiarazione di voto per cercare di fare un po' di chiarezza sull'oggetto della discussione di queste ultime ore, di ieri sera e di questa mattina. Ho sentito questa mattina il presidente Quagliariello dire con assoluta tranquillità che, a suo giudizio, sul punto che riguarda lo stato giuridico dei professori e dei ricercatori di ruolo, la volontà del legislatore così come emerge da questa legge

«fatto salvo», perché scrive un comma 4 del tutto aggiuntivo, che possiamo leggere, in cui si dice, modificando il testo del comma 11 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005, che a a questi dipendenti pubblici «è attribuito il titolo di professore aggregato per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi e moduli. Il titolo è conservato altresì nei periodi di congedo straordinario per motivi di studio di cui il ricercatore usufruisce nell'anno successivo a quello in cui ha svolto tali corsi e moduli». Quindi, la Camera dei deputati non vuole fare salvo quanto è previsto dal comma 11 dell'articolo 1 della legge in questione, ma modificarlo nel senso di consentire l'uso del titolo di professore aggregato

Per cui, dopo aver stabilito che quel titolo si conserva anche nell'anno successivo a quello in cui si sono svolti i corsi, modifica il comma 11 dell'articolo 1 della legge n. 230 del 2005 e che in quel comma non deve essere scritto «per il periodo di durata degli stessi corsi e moduli» - ossia un periodo molto più corto - bensì

Se la legge si fermasse a questo punto, la volontà del legislatore sarebbe assolutamente chiara: non vogliamo abrogare quanto è previsto dal comma 11 dell'articolo 1 della legge n. 230, ma vogliamo modificarlo nel senso di consentire l'uso di quel titolo, cioè professore aggregato, a condizioni diverse da quelle previste dal comma. È però del tutto evidente che se nella stessa legge si interviene abrogando - come fa l'articolo 29 - il comma 11 nel suo complesso, si ha una legge nella quale la volontà del legislatore è

consente a coloro che lo vogliono usare nell'anno accademico in cui hanno svolto quel corso? Solo nel momento in cui c'è il corso possono usufruire di quel titolo, o addirittura nell'anno successivo a quello in cui hanno fatto il corso? Sono tre soluzioni tra di loro diverse che a questo punto, sulla base di detta legge, sono legislazione vigente. Ora mi dica lei, signor Presidente, se non sia razionale sostenere che il Presidente del Senato debba ordinare le votazioni in modo tale che questa Aula non decida sulla stessa questione

Pensate che si possa fare un decreto successivo, dopo la promulgazione della legge, che consenta di sanare un'operazione di questo tipo, quando la sanatoria si può realizzare - udite, udite - rimandando alla Camera questo testo di legge

della promulgazione della norma. In caso contrario, è in vigore una norma che non consente a nessuno di sapere chi si può fregiare del titolo di professore aggregato e in quali condizioni. E questo, solo perché avete paura,

partecipo al dibattito politico del Paese, in realtà, sulla base di questo presupposto. Ma se voi oggi date questo spettacolo (il Regolamento qui non c'entra), è perché avete addirittura paura della vostra ombra: alla Camera dei deputati non ci si può più andare nemmeno per togliere la parola «11» da una legge e state dicendo che farete PD e IdV).* Dal punto di vista politico dimostrate di non avere alcuna forza e capacità di orientamento

Signora Ministro, l'articolo 10 ha ad oggetto la competenza disciplinare

è oggettivamente incomprensibile, perché già le sanzioni vengono proposte da organi al cui interno gli studenti non sono presenti e - quindi - non capiamo perché l'organo che dovrà definire la sanzione al termine di questo procedimento debba essere solo parziale e non completo. Credo che dopo l'immagine che questo Senato ha dato ieri, dopo la volontà precisa da parte del Ministero di non comunicare con gli studenti e di non volere un colloquio vero, reale, fattivo

D'altra parte tutti, chi più chi meno, riteniamo che la partecipazione degli studenti sia importante nell'esprimere un contributo a giudicare la qualità dell'insegnamento. Sono state trovate varie forme interlocutorie, quiz, sedute, scritti, interlocuzioni. Gli studenti dunque hanno ormai, per volontà comune, il diritto di esprimere opinioni sulla qualità dell'insegnamento che ricevono. È del tutto illogico che gli studenti cui si riconosce questo diritto non possano contribuire in modo assolutamente minoritario ad una decisione sulle questioni di disciplina. Non c'è razionalità in questa misura e non c'è nemmeno rispetto della verità e della realtà: siamo fuori da una logica Non si capisce perché gli studenti non debbano essere presenti quando sul resto della vita universitaria possono fornire opinioni, indirizzi e progettualità.

nelle università e negli organismi di rappresentanza, questo è davvero un atto inspiegabile e quindi preannuncio parere contrario

una concezione autoritaria e non partecipativa e quindi gli studenti non possono essere parte di un collegio. Invito dunque ad accogliere il nostro intervento emendativo che corregge una stortura.

*(FLI)*. Signor Presidente, dichiaro il mio voto di astensione sui due emendamenti 10.1 e 10.2, perché condivido l'assoluta necessità della partecipazione degli studenti, ma c'è un tema a monte che vorrei sollevare: qual è la partecipazione degli studenti oggi nell'università italiana? Un esiguo numero di studenti frequenta l'università rispetto al totale degli iscritti, e questo è un gravissimo *vulnus*, che non avviene in alcuna università civile del mondo. Un ulteriore esiguo numero di studenti che frequentano, partecipa alle elezioni e quindi alla rappresentanza. E quindi, quale rappresentanza rappresentano coloro che rappresentano gli studenti? Questo è il tema vero. E se posso permettermi da quest'Aula un suggerimento agli studenti che vogliono protestare liberamente, la vera forma di protesta che metterebbe in difficoltà l'intera classe dirigente italiana e questo Parlamento sarebbe concordare, una mattina alle ore 9, la presenza di tutti gli iscritti all'università nelle aule universitarie: toccheremmo con mano che esploderebbero. Ci sono facoltà con 25.000 iscritti per esperienza personale - e 3.000-4.000 frequentanti. L'intera struttura è tarata sui 25.000 iscritti e poi ci troviamo un docente per ogni 4 studenti effettivamente frequentanti. Per questo mi asterrò

Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento. Le faccio notare, ancora una volta, che il testo pervenuto dalla Camera presenta incongruità veramente eccezionali: non ho mai visto una cosa del genere. Infatti, mentre nell'articolo 10, al comma 1, si parla dell'istituzione del collegio di disciplina composto esclusivamente da professori universitari in regime a tempo pieno e ricercatori a tempo indeterminato in regime a tempo pieno, pieno, passando alla possibilità, capacità e potestà di infliggere una punizione si vengono ad escludere gli studenti come rappresentanza dentro un consiglio d'amministrazione che invece li prevede.

se una realtà come quella studentesca fa parte del consiglio d'amministrazione non si vede perché, nel momento in cui trattasi di infliggere una sanzione, peraltro già comminata da quello che è il collegio di disciplina, debbano essere estromessi proprio gli studenti, che sono *pars* attiva e *costruens* di tutto il sistema universitario, insieme ai professori ed al personale non docente. O è una comunità o non è una comunità. E siccome la logica disciplinare intende anche prendere in considerazione, Presidente, la comunità ed il contesto in cui una violazione è stata consumata, credo sia assolutamente inconcepibile prevedere che gli studenti possano non far parte

altresì sottolineare ai Sottosegretari che sono qui presenti che quello che colpisce molto in questo disegno di legge è l'assenza della figura degli studenti. Stiamo parlando dell'università dal punto di vista della *governance*, dal punto di vista dei docenti e mai vi è la figura degli studenti. Pensate, ad esempio, come abbiamo discusso sul diritto allo studio: c'è una delega: punto e basta, senza alcuna indicazione di criteri, di direttive o di obiettivi. Abbiamo persino rifiutato di sottolineare l'importanza, all'interno del diritto allo studio, degli studenti disabili, ai quali non è consentito molto spesso, a causa delle barriere architettoniche o della mancanza di strumentazioni didattiche, di partecipare all'attività e ai corsi universitari. Qui abbiamo la emblematizzazione dell'assenza degli studenti: eliminiamo

organo non può essere composto ad elastico, aumentandolo o riducendolo a seconda delle determinazioni che vengono fatte se non sulla base di criteri, che sono ad esempio gli elementi di incompatibilità

con la sottolineatura quindi che gli studenti non sono per nulla presenti all'interno di questo disegno di legge, ma anche dal punto di vista giuridico e istituzionale. Siamo davvero all'interno di una inaccettabilità ma anche irragionevolezza di questo testo. Quindi, non solo dichiaro il nostro voto favorevole, ma chiedo davvero di porgere un'attenzione particolare a questo emendamento, accettando l'introduzione della parola «con» in sostituzione della parola

all'emendamento. Poi, ovviamente, sono costretta a parlare in dissenso dal Gruppo perché trovo troppo moderate le parole che ha usato la senatrice che ha usato la senatrice Bastico per sostenere queste ragioni. Io invito il Ministro - che purtroppo non vedo - visto che farà il decreto per correggere l'articolo 5, di correggere anche questo, perché è un'altro punto di dubbia costituzionalità oltre che essere un messaggio che è peggio che criminalizzante nei confronti degli studenti. Li si considera dei minori,

possono votare, eleggere tutti noi e non possono votare in un organo collegiale se il provvedimento è disciplinare? È questo il conflitto d'interesse che avete in mente, signori? Pensateci, perché è un grande errore quello che state facendo!

è l'estrema difesa sull'argomento che abbiamo sostenuto fino ad adesso, anche con il contributo dei colleghi del Partito Democratico. Bocciati gli emendamenti precedenti, era una maniera per provare a sanare il danno. Questo emendamento deve fronteggiare l'obiezione del collega Baldassarri, che non manca di una sua dignità sociologica. È vero che gli studenti non partecipano agli organismi di rappresentanza. È vero che gli studenti votano poco e che le rappresentanze ufficiali degli studenti sono ridotte*. Questo è un problema che il Parlamento dovrebbe considerare con maggiore serietà. È veramente curioso che fronteggi questo, che dovrebbe essere un problema di inclusione, con una logica di esclusione. Siccome non partecipano tanto vale farli fuori dalle commissioni che stabiliscono i provvedimenti disciplinari. dovrebbero trovare nel Parlamento una leva persuasiva per essere convinti a dare un contributo costruttivo, quindi anche negli organismi ufficiali. In questa maniera non lo si fa: non credo che si potranno persuadere gli studenti a partecipare agli organi istituzionali tramite la graziosa regola per cui loro devono stare fuori. È veramente una cosa che sembra straordinariamente incoerente.

voglio motivare molto brevemente. In un momento così teso - non voglio dire drammatico - in cui ci rivolgiamo agli studenti e cerchiamo di riportare tutto in una condizione di legalità, e su questo abbiamo anche dei segnali rilevanti da parte del movimento studentesco, noi votiamo queste norme che escludono in maniera incomprensibile oltre che incostituzionale la partecipazione ad un organismo che deve giudicare gli studenti: escludiamo la loro componente dopo battaglie di decenni per integrare questi organismi rappresentativi. Per questi motivi, mi astengo dal voto

l'uno, abbastanza sottolineato dai miei colleghi, con l'espressione «senza la rappresentanza degli studenti»; e l'altro con il termine «vincolante», che è assolutamente pleonastico in quanto già il testo precedentemente diceva «conformemente al parere espresso dal collegio di disciplina» e quindi è assolutamente inutile. La cosa che sconvolge, però, è questa previsione: «senza la rappresentanza degli studenti». Non ripeterò le cose che hanno detto esplicitamente i colleghi, però chiedo agli amici di buon senso di quest'Aula, innanzi tutto ai colleghi della maggioranza: quale può essere la *ratio* di questa norma? norma? Non si riesce a comprendere. Se si va all'articolo 2 che prevede la composizione del consiglio di amministrazione, signor Presidente, si legge che l'unica rappresentanza elettiva - l'unica: le altre sono o di diritto o designate o scelte - è quella degli studenti. Gli studenti che sono parte del consiglio di amministrazione sono quelli che realmente rappresentano gli studenti dell'università.

Quale può essere la *ratio* di un'esclusione di questo genere? dei senatori qui presenti, compresi i senatori di maggioranza, sono intimamente contrari a questa norma perché non c'è nemmeno la capacità di spiegarla. Sarei veramente curioso di sentire qual è la *ratio* che la disciplina. Quando - se andrete - ad inserirla in sede di conversione del decreto milleproroghe in una data sicuramente più tarda rispetto a quella di un passaggio veloce alla Camera. Signor Presidente, stiamo compiendo delle storture che nessuno vuole, nemmeno gli amici della maggioranza, perché siamo costretti dai tempi. Cerchiamo di dare un minimo di respiro a quest'Aula e a questa riforma. Non ci sono scadenze. Noi siamo anche disponibili a tornare in Commissione, con un lavoro coordinato, affinché si arrivi

una diffidenza di fondo nei confronti della soggettività e della personalità degli studenti. Signora Ministro, vorrei dirle che non si potrà mai costruire un'università forte ed autorevole senza la presa di posizione, la consapevolezza, la decisione e la partecipazione degli studenti.

della rappresentanza, come ha ricordato anche il collega Di Giovan Paolo. Sulla rappresentanza si fa la nuova classe dirigente. Lo abbiamo fatto noi, fatelo anche voi, ma non tappate la bocca, perché sa tanto di ritorno al fascismo.

confligge con il buonsenso, con l'opportunità dei tempi e con la storia democratica di partecipazione, nella quale credo ci siamo formati *bipartisan* nelle università e nei licei.

che ritengo assolutamente contrario alla dignità degli studenti. A tale riguardo, vorrei ricordare che molto spesso si parla

attraverso la presenza di commilitoni che possano valutare questo particolare aspetto.

debbo sottolineare al Ministro che autonomia (soprattutto nell'università, ma comunque sempre nel settore scolastico) significa una cosa sola: responsabilità diffusa,

dell'università stessa, cioè lo studente. Lo studente ha il diritto di essere compreso, ricompreso e protagonista di tutti i processi

lesiva dell'autonomia universitaria, perché viene a mancare la parte più significativa e delicata che è appunto il collegio degli studenti e, quindi, la presenza degli studenti negli organismi *(PdL)*. Signor Presidente, signore e signori del Senato, io amo molto la demagogia

10, ho sentito affermazioni che non sono assolutamente corrispondenti alla realtà normativa. Innanzitutto, la competenza disciplinare dell'articolo 10 prevista esclusivamente per il professore o il ricercatore sottoposto ad azione disciplinare. Cari colleghi, qui non si giudicano gli studenti: si giudicano soltanto i professori o i ricercatori. Il collegio di disciplina è infatti composto esclusivamente da professori universitari in regime di tempo pieno e da ricercatori a tempo indeterminato; essi giudicano esclusivamente sugli eventuali illeciti disciplinari di professori o di ricercatori, non degli

semplicemente esecutivo di quello che decide nell'*an* e nel *quantum* il collegio di disciplina. Quindi la partecipazione degli studenti, che ci sia o non ci sia, è assolutamente indifferente. *(Commenti della senatrice Adamo).* È azzerato il potere del consiglio d'amministrazione, il quale prende atto semplicemente di quello che ha deciso il collegio di disciplina. Questa è la realtà. Allora, se vogliamo difendere il consiglio d'amministrazione, dobbiamo difenderlo tutto, dicendo che non solo devono esserci gli studenti, ma anche che devono esprimere il loro parere su quello che è stato già detto essere un parere vincolante nell'*an* e nel *quantum*. *(Applausi dal Signor Presidente, non parteciperò al voto sull'articolo 10 per non essere in alcun modo corresponsabile di una scelta che nega la storia stessa delle università e in particolare delle università italiane che sono nate molti secoli fa come comunità di studenti, che spesso avevano anche il potere di sanzionare i professori che venivano meno ai loro doveri e ai loro compiti. Rovesciare la storia delle università italiane sulla base di una visione effettivamente un po' fascista, ma anche di strettissima prospettiva, significa davvero condannare il nostro sistema universitario all'assenza non solo di passato ma anche di futuro. Per non essere

di collaborazione con gli studenti impegnati appunto nei luoghi della decisione, peraltro con difficoltà sempre fortissime. Ho visto crescere quei ragazzi e li ho visti diventare non solo degli ottimi professionisti, ma anche persone che si sanno occupare degli altri e che sono cresciuti con la politica dall'università nella società.

Signor Presidente, mi trovo nella necessità di ricorrere a questo strumento d'Aula per poter azzardare una risposta a quanti hanno ritenuto di poterci bollare come populisti nel momento in cui hanno preso atto delle nostre dichiarazioni. La verità è che questa gioventù è già stata espropriata del proprio futuro. Con comportamenti come quello che si vorrebbe realizzare con questo provvedimento, si vorrebbe anche commissariare l'intelligenza, si vorrebbe cioè affermare che ai giovani, in ragione della loro condizione, non può essere concessa la facoltà di svolgere un ruolo attivo nella loro università.

la sospensione del giudizio nel caso di rinnovo del consiglio d'amministrazione. Siccome noi sappiamo che il consiglio d'amministrazione può anche essere rinnovato in tempi differenti, si arriva al paradosso di poter sospendere il giudizio in attesa del rinnovo, per esempio, proprio della componente studentesca che poi viene esclusa dalla possibilità

Quindi, per senso di responsabilità, ovviamente, condividendo l'impianto complessivo della legge, noi comunque votiamo a favore di questo articolo 10, ma con un invito al Ministro perché nei decreti attuativi possa, in qualche modo, proseguire il discorso iniziato al Senato e, in qualche modo, annacquato alla Camera.

Smettetela di dire bugie e falsità! Siete degli irresponsabili! che noi sputiamo in faccia agli studenti, rispondo che siete voi che in questo momento lo state facendo! Noi abbiamo rispetto per gli studenti. Abbiamo tanto rispetto da non dire le bugie e le falsità che state dicendo voi in Aula in questo momento!

rivolti all'opposizione lui non se li può permettere! Ieri quest'Aula è stata teatro di decisioni inaccettabili, che hanno modificato fortemente i modi di stare in Aula e che influiranno sul futuro di questa legislatura. La responsabilità di quel che è successo ieri grava tutta sulle spalle del Vice Presidente che ieri presiedeva l'Aula mi dispiace dirlo, signor Presidente, per le sue successive decisioni che noi tutt'ora non condividiamo. A questo punto, lei convochi la Conferenza dei Capigruppo, alla quale io assumere decisioni equilibrate, che tengano conto della sostanza della questione e degli equilibri d'Aula, ma invito il senatore Bricolo a legarsi la lingua quando parla *(Proteste dal Gruppo LNP)*, perché non può parlare di noi in questo modo!

dell'Assemblea è rimasto immutato e i lavori proseguono ad oltranza fino a quando non finiremo di lavorare.

«può, su proposta dell'ANVUR, essere ridotto». La cosa ha un significato preciso. L'ANVUR è il grande fantasma di questo disegno

la possibilità di stabilire una prassi di valutazione, ma questo organo, che dovrebbe garantire la prassi di valutazione, è ancora nel regno del nulla.

al fine di vedere se davvero quest'organo di valutazione può essere saggiato sull'insieme degli argomenti a proposito dei quali è legittimo aspettarsi che si debba pronunciare. Quindi, consideriamo molto importante questo emendamento, nient'affatto di maniera, perché è uno stimolo anche costruttivo a garantire che la prassi di valutazione venga finalmente materializzata e realizzata. materializzata e realizzata.

alle vicende che si sono snodate tra ieri pomeriggio e stamattina abbiamo fatto un'offerta alla maggioranza, alla Presidenza del Senato e al ministro Noi abbiamo posto una questione, che attiene alla regolarità del procedimento legislativo e alla difesa dell'autonomia delle prerogative del Senato rispetto al Governo di legge che non ha nessuna data di scadenza, nessun termine perentorio da osservare; questo provvedimento infatti non è né una legge finanziaria né una legge di stabilità né un documento che debba essere approvato entro un termine certo. Abbiamo detto: ci sia l'intesa per eliminare dal testo l'articolo 29 e non tornare ad ulteriori due deliberazioni affermative di quell'articolo 29, che poi si delegherebbe il Governo ad eliminare con un provvedimento successivo di qualsiasi e l'esame del testo verrà concluso regolarmente, con i tempi utili a discutere ma senza alcuna ulteriore remora di natura strumentale. Di fronte a questa, secondo me, ragionevolissima proposta, che tiene conto non del merito del provvedimento - rispetto al quale eravamo e restiamo contrari ma delle prerogative del Senato e della correttezza del procedimento legislativo, ci è stato risposto in maniera negativa. A questo punto, il mio Gruppo non ritiene di accedere a nessun accordo sul prosieguo dei lavori. Ciascuno si assumerà la sua responsabilità, ovviamente. Noi abbiamo assicurato che la nostra presenza in quest'Aula sarà connotata dalla possibilità di fare ricorso ad ogni strumento previsto dal Regolamento ma senza intenzione di incendiare alcunché.

non mettere paletti nel corso dei lavori. Conosciamo il nostro ruolo, abbiamo sottolineato quello che nelle procedure non ci ha convinto perché è sbagliato, vogliamo essere in Aula garantendo la nostra presenza a discutere nelle forme che il Regolamento parlamentare ha consacrato.

al quale chiedo anche di aggiungere la firma, desidero semplicemente sottolineare con assoluta necessità che noi qui sentiamo la differenza, lavorando nel merito in questo caso, tra la serietà e la distrazione. All'articolo 11 si parla degli interventi perequativi sui finanziamenti alle università statali secondo la misura della qualità.

ma attiene a maggior ragione in Parlamento ai Gruppi di maggioranza e di opposizione che sono qui per fare esattamente questo mestiere, in nome del popolo italiano, usando non la sciatteria, ma la serietà.

questo emendamento ci pone di fronte, non per la prima né per l'ultima volta, ad un tema di qualità legislativa.

nella dimensione legislativa una sorta di libertà di interpretazione e si annulla la possibilità di

la consegna di una sorta di arbitrarietà alle autorità che se ne devono occupare e, nello stesso tempo, è in contrasto intimo con la vocazione che questo provvedimento mostra, soprattutto in tutte quelle aggiunte correttive che la Camera ha introdotto nel testo.

Invece, soprattutto gli inserimenti della Camera insistono nella proliferazione di una sorta di voluttà della ridondanza normatrice, con un eccesso di precisazioni, cavilli e indicazioni

appesantisce e rende vacuo il testo.

ovviamente ho preso atto della dichiarazione di inammissibilità dell'emendamento 11.300, e non ho titolo per contestare tale giudizio. Tuttavia, questo emendamento,

atenei, poiché, in base ai criteri di valutazione adottati, si determinano esiti assolutamente dannosi per quelle areeterritoriali che vivono condizioni economico‑sociali profondamente diversificate. Per esempio, l'anno scorso, uno degli elementi di valutazione era quello legato al numero dei laureati assunti nel sistema industriale di riferimento regionale. Capite bene che un criterio di questo tipo determina una

Se ci fosse una legge elettorale diversa e gli eletti dovessero rispondere agli elettori, e non soltanto a chi li porta in Parlamento (tutti noi siamo stati trasportati o paracadutati in Parlamento, e invece sarebbe preferibile che i parlamentari derivassero il loro titolo

evidente, infatti, che i sistemi industriali e socio‑economici del Mezzogiorno sono molto più deboli di quelli settentrionali e quindi i termini di valutazione sono assolutamente ingiusti. generico, se volete - era un'indicazione programmatica perché ci fosse una ponderazione di queste condizioni e venisse consentito anche alle università meridionali, che sono impegnate in sforzi di razionalizzazione onerosissimi proprio per le loro condizioni di difficoltà economiche, di avere appunto degli interventi di aggiustamento e di ponderazione che attutiscano questi effetti così gravi. Al di là dell'inammissibilità tecnica dell'emendamento, non contavo in alcun modo sul fatto che vi fosse un apprezzamento politico da parte della maggioranza e del Governo, non solo per questa maledetta blindatura del testo che ci sta regalando una sessione parlamentare imbarazzante, per cui ci si rifiuta di cogliere anche delle difformità e delle disomogeneità formali,

Al di là del fatto che la blindatura rendeva impossibile l'accoglimento e al di là dell'inammissibilità, c'è una indisponibilità culturale di questo Governo, al di là della retorica, dei piani per il Sud e di tutte le costruzioni artificiose, che è anche di ordine politico, come dimostra il fatto che ci si sta apprestando nell'area di maggioranza per imbrogliare ancora una volta l'elettorato meridionale, cercando di nascondere che questo Governo è allocato non solo geograficamente, ma intellettualmente, socialmente ed economicamente nel Nord. Nord. Questa è la sostanza. Ieri, il ministro Gelmini, in modo non dico improvvido ma onesto, riteneva che fosse naturale che i tagli sui fondi ordinari per il diritto allo studio fossero coperti attraverso il piano per il Sud, che è alimentato dai fondi strutturali e per le politiche di coesione. Anche in questo caso, questa costruzione risente di un difetto di un difetto d'origine per cui non si riconosce alcuna valenza, alcuna responsabilità al Governo di farsi carico di una politica di riequilibrio e di coesione, mentre è responsabile di una politica che sta allargando il divario, sta penalizzando il Mezzogiorno e lo sta impoverendo in modo drammatico.

come titolo «Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario». Non so se sia una sorta di nemesi che un provvedimento di questo tipo contenga tali e tanti errori giuridici, materiali, articoli che ne contraddicono altri, da non consentire davvero anche ad uno studente del primo anno di giurisprudenza di promuoverne il testo. Signor Presidente, le modifiche apportate dall'altro ramo del Parlamento all'articolo 11 introducono, nel calcolo degli squilibri finanziari dei singoli atenei, la specificità delle università sede di facoltà di medicina e chirurgia collegate ad aziende ospedaliere nate da ex policlinici a gestione diretta,

medesimo articolo, la ripartizione della percentuale indicata nel comma 1 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Il mio Gruppo ha annunciato il voto contrario all'articolo 11, il quale meriterebbe un approfondimento sostanziale. Si tratta anche di valutare le modifiche introdotte nell'altro ramo del Parlamento, ma purtroppo la maggioranza è sorda e cieca e in quest'Aula non permette il dibattito, avendo blindato di fatto questo provvedimento. Termino, signor Presidente, perché

la maggioranza è sorda, non vede quello che accade fuori di qui. Non vogliamo fomentare alcuna rivolta, vogliamo solo rispettare coloro che hanno diritto a manifestare pacificamente, mentre prendiamo le distanze dai violenti. Per questa ragione, signor Presidente, la maggioranza non ci permette di dibattere, ha blindato questo provvedimento e, dato che non sono convinto della bontà dell'andamento dei lavori di questa Aula e non intendo votare contro questo articolo, annuncio il

si dice che l'intervento perequativo deve essere ridotto proporzionalmente se la situazione di sottofinanziamento deriva da una valutazione negativa della qualità non può che essere l'ANVUR

alla logica che cerca di mortificare sempre più gli atenei già in difficoltà. Vorrei soltanto ricordare che prima di questa riforma sono stati praticati

dico rivolgendomi soprattutto ai colleghi della Lega - un federalismo reale, soprattutto se l'emendamento del collega Pistorio fosse stato tenuto in buon conto. Il federalismo non è solo dato dalle autonomie locali: è un sistema e un metodo e l'unico federalismo è il federalismo solidale. La verità è che votando questo articolo la maggioranza e la Lega inaugurano un nuovo tipo di federalismo, un federalismo borghese che potremmo definire *federal chic.* Presidente, con estremo rammarico sono costretto ad esprimere il mio dissenso dalla posizione del Gruppo in quanto, a mio avviso, non è stata sottolineata adeguamento l'aleatorietà di questo articolo che poi sostanzialmente descrive l'aleatorietà dell'intero impianto del provvedimento che attualmente stiamo votando. Infatti, già al primo comma,

non statali. Entro nel merito rivolgendomi al Ministro per dire che la situazione di oggi è radicalmente diversa rispetto a quella degli anni '50. Personalmente ritengo che un Paese civile, che vuole competere in termini di conoscenza, abbia bisogno di una solida e ben strutturata università statale e abbia altrettanto bisogno di una solida e creativa università libera.

Ebbene, la perequazione viene operata quando c'è divario, sperequazione, ma questo articolo non determina le modalità per misurare la sperequazione e non mette in campo neppure gli strumenti per contemperare la sperequazione determinata da deficit

che devono misurare il merito di ciascuna istituzione universitaria. Trovo che con questa previsione le istituzioni universitarie che vivono già situazioni di difficoltà non potranno porsi l'obiettivo di migliorare la propria qualità, perché mancheranno le risorse per garantire quegli investimenti necessari a determinare una nuova fase misurabile in termini di efficienza.

*(IdV)*. Nel cappello introduttivo di questo articolo si legge: «Al fine di incentivare la correlazione tra la distribuzione delle risorse statali e il conseguimento di risultati di particolare rilievo nel campo della didattica e della ricerca (...)». Questo articolo, quindi, è in assoluta armonia con quello che

e all'efficienza del sistema universitario, e introdurre meccanismi premiali anche nella distribuzione delle risorse pubbliche. Allora, se è vero - come ci ha spiegato il Governo - che questo è lo spirito della legge, se è vero che il dato letterale che ho appena letto all'Aula va in questa direzione,

che cosa si vuole derogare per le università telematiche. Si vuole derogare ai criteri di distribuzione delle risorse pubbliche? Si vuole derogare alla necessità di avere un sistema che vada nella direzione della qualità e dell'efficienza del servizio universitario fornito? Non si capisce. Questa deroga non ci convince.

in merito alla vicenda del CEPU, che qualcuno ha voluto collegare con il voto di sfiducia alla Camera. Non intendo farlo, perché lei ha già presentato in Aula in via preventiva le sue argomentazioni. D'altra parte, noi abbiamo approfondito molto questo tema in Commissione, per cui, lungi da me detto argomento.

12.3. Forse è l'unico modo per escludere qualsiasi cattivo pensiero intorno a questo elemento. Noi proponiamo di cancellare dal comma 3 dell'articolo 12 dalle parole: «ad eccezione di quelle» fino alla fine

introdurre una qualche riduzione del danno. Ma questa riduzione del danno è, a nostro avviso, assolutamente inadeguata, perché le caratteristiche per l'accesso da parte delle università telematiche verranno individuate con decreto del Ministro, sentita l'ANVUR. Non cioè, alcun vincolo del parere dell'ANVUR e - quindi - nessuna garanzia di terzietà rispetto a tali valutazioni. I criteri a cui si rinvia sono quelli del comma precedente, che per altro stabilisce dei criteri molto, ma molto labili. Pertanto la richiesta - molto sentita rivolgo a tutti è fatta per amore di verità (prima il presidente Possa mi ha invitato in tal senso): facciamolo per amore di verità, togliamo tutta questa parte, togliamo qualsiasi possibilità di interpretazione e di lettura e stabiliamo semplicemente che le università telematiche non possono accedere

Le 11 università telematiche forse andrebbero in gran parte chiuse e non rese destinatarie di fondi pubblici. Basta che il ministro Gelmini legga il rapporto del Comitato nazionale sul sistema universitario per vedere come, nel capitolo 7, vengono valutate le nostre università telematiche: non hanno docenti, hanno studenti fittizi e hanno un'enormità di programmi di studio e corsi di laurea, c'è stata una proliferazione di questa istituzione. Bisognerebbe allora essere molto cauti nel decretare

vuoto legislativo e pertanto dichiariamo il nostro voto contrario e vorrei far riflettere anche altri componenti del Gruppo dell'Italia dei Valori sull'opportunità di esprimersi in modo analogo al Partito Democratico.

almeno per una questione di dignità di tutte le università e delle persone serie che lavorano all'interno delle università, possiamo dire che le università informatiche sono un non senso? Almeno questo lo dichiariamo anche ai giovani che stanno manifestando fuori? Signora Ministro, mi auguro che anche lei, nella difesa della qualità della nostra università, dichiari, senza se

Diciamolo con chiarezza, soprattutto per chi qui ha figli e nipoti, che magari in questo momento stanno frequentando con dignità l'università, come la sottoscritta! Credo che dobbiamo lanciare all'esterno un messaggio chiaro ed inequivocabile su questo punto! chiedo al Ministro di dire con chiarezza il senso di questo comma, perché così com'è è senza senso. Almeno, io non ne ho capito il senso e desidererei capirlo. *(Applausi dal Gruppo

meglio la nascita, la gestione ed il governo delle università telematiche. Infatti, come ha detto la senatrice Baio, mentre il testo viene presentato come la *summa* della difesa della serietà e della severità degli studi universitari, questo comma introdotto alla Camera apre una vulnerabilità dei principi che vengono propagandati e che accompagnano il testo di legge. Per questa ragione, mi asterrò dal voto.

ha ridotto la discussione ad un problema di ordine pubblico, non ha capito che il movimento degli studenti ha ragioni profonde. È il sintomo preoccupante di una generazione che non ha futuro, senatore Quagliariello: non ha futuro, le abbiamo rubato il futuro, tutti. Ragazzi allibiti dalla politica, che raccontano ai giornali di essere angosciati dalla disoccupazione, dalla prospettiva del lavoro che manca.

Gasparri! Gli studenti non rimarranno a casa, perché l'università è la loro casa, ma non cadranno neppure nella trappola di farsi passare per violenti: gli studenti, questa generazione, ha tutti i diritti, come la

una comune maniera di stare nella maggioranza con il formando terzo polo, che poi invece ha votato la sfiducia a questo Governo ed a questa maggioranza. Quindi, l'emendamento si è trasformato in quel momento da «polo d'oro» in «Polidori», in quanto l'unica benefattrice di questo*...

Signor Presidente, con pacatezza, ma anche con fermezza, desidererei entrare nel merito della questione. Credo che questo comma 3 aggiunto dalla Camera dei deputati

scarsissimi fondi disponibili tra le università statali e non statali. *Nulla quaestio*, perché facciamo riferimento comunque a dei parametri ben individuati ed identificati, che dovrebbero attestare comunque la situazione di fatto in cui versano queste università non statali, meritevole di avere questo tipo di contributo, peraltro aumentato di 10 punti (dal 10 per cento siamo passati al 20). Ma che poi si dica che si dica che la previsione di quest'articolo, vale a dire della distribuzione dei fondi, non si applica alle università telematiche ad eccezione di quelle individuate con decreto del Ministro, e così è veramente una cosa non accettabile. Vede, Ministro: siamo ancora in una fase in cui lei non ha nessuna capacità né esistono atti di merito con i quali poter valutare l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza, la consistenza e la serietà di questo tipo di università, che potranno anche essere benemerite: non faccio né il processo alle intenzioni né voglio mettere il carro davanti ai buoi. Ma certamente sta di fatto che se agiamo con assoluto rigore rispetto alla spartizione di una torta, che è il fondo per le università, per il merito e per tutto quello che ne consegue che riguarda le università statali e quelle non statali legalmente riconosciute, non possiamo però aprire i cordoni di una borsa così stretta e così misera semplicemente con l'individuazione di un decreto da parte sua, che non fa riferimento a nessun tipo di parametro di valutazione, a nessun sistema di controllo, a nessun sistema di verifica acclarata. Lasciarsi prendere dal modernismo può essere anche un grave difetto. Parlare di modernizzazione è qualcosa di molto serio: significa accogliere anche le istanze che provengono dalla società, dal mondo scientifico ed accademico, che possono aprire anche degli squarci di prospettiva in mondi che non sono stereotipi, secondo la cultura tradizionale. Quindi, perché no, anche l'università telematica. Non metto il carro davanti ai buoi, ma che ci siano un controllo, parametri certi, criteri condivisi e non sia tutto dato alla discrezione del Ministro, sentito un parere che non è neanche vincolante per la distribuzione di scarsissime risorse che spetterebbero innanzitutto alle università statali, mi sembra veramente troppo. Quindi condividiamo questi emendamenti e chiediamo di apporvi la nostra firma.

molto del lavoro che facciamo insieme in quest'Aula, però vorrei intervenire in dissenso per dire una cosa. Noi sappiamo che siamo in un quadro di decurtazione perché, assunto il contributo alle scuole non statali, di questo 100 il 20 va solo sulla base della qualità. E questo è un principio che noi sosteniamo, sapendo però che non stiamo dando incentivi alla qualità: stiamo sottraendo prima il finanziamento ordinario e poi lo diamo, ma solo sulla base degli incentivi. A questo punto, però, definendo il fondo come fondo della qualità,

ha interrotto la senatrice Adamo: non si fa. Comunque, io penso che equiparare le università telematiche ad università come la Bocconi e altre private sia un delitto. cosa serve? Non voglio pensare alla Camera: quando mai? Siete uomini d'onore, direbbe Shakespeare! Penso alla pubblicità, ai cartelloni, ai divi del calcio che fanno pubblicità a cose inesistenti.

in questo momento la circostanza, ma nel momento in cui si parla di una riforma dell'università ci sono delle priorità, e le priorità, quando si tagliano le risorse, devono riguardare innanzi tutto le realtà che esistono, che funzionano e che sono rodate, e quindi le università statali.

Stavo dicendo che quando si fa una riforma universitaria, e la si fa avendo come presupposto un taglio consistente delle risorse all'università, si fanno delle scelte e si individuano delle priorità. Le scelte e le priorità riguardano evidentemente quelle realtà che esistono, che funzionano, che hanno una serie di problemi; e tra queste, ovviamente, le priorità non possono che riguardare in via esclusiva le università statali e non statali che hanno una loro tradizione accademica e un loro radicamento, offrono la qualità di un servizio, fanno ricerca, e via dicendo. Ora, il mondo delle università telematiche sarà certamente il il mondo del futuro, sarà il nuovo modo di apprendere e di studiare; ad oggi, senza voler nulla togliere a chi fa questo lavoro, in in parecchie circostanze ci è capitato di vedere neolaureati in avanzato stato di età che si sono

non sia in linea e contraddica lo spirito di una riforma che vuole puntare sulla qualità e sull'efficienza e che punta peraltro a ridurre nel tempo - almeno così leggo nell'idea del federalismo universitario - anche le sedi universitarie, un tema questo estremamente importante. La cosa che ulteriormente ci lascia molto, ma molto perplessi è anche la circostanza che, con tutto il rispetto nei confronti della signora Ministro, si prevede di individuare con un decreto discrezionale le università telematiche che possono accedere a quei fondi

all'esclusivo potere discrezionale del Ministro la scelta e la selezione di queste università, come pure il trasferimento dei fondi. Quindi, al di là lei retropensieri e dei processi alle intenzioni, che nessuno qui vuole fare, credo che questa norma sia obiettivamente scandalosa e che vulneri i princìpi della riforma universitaria, che puntano a selezionare le università, a ridurne nel tempo il numero e a concentrare le risorse su quelle che dimostrino di svolgere il lavoro con dedizione, indipendentemente dal fatto che siano pubbliche o private perché, dal nostro punto di vista, ciò che è pubblico è il servizio che viene reso e non il soggetto che lo rende. dunque che sia obiettivamente un fuor d'opera, una contraddizione e che sia peraltro troppo ampio il margine che viene concesso al Ministro di scegliere,

Signor Presidente, in data 8 aprile 2009 scrissi al presidente Schifani una lettera per proporgli di integrare la cosiddetta galleria dei Presidenti, alle spalle dell'Aula del Senato, con il ritratto del senatore Giovanni Spagnolli, che fu Presidente del Senato della Repubblica dal giugno 1973 al luglio 1976 e del quale nel 2009 ricorrevano i 25 anni dalla morte. Mi onoro di rappresentare in quest'Aula lo stesso collegio elettorale del senatore Spagnolli, quello di Rovereto. In data 22 aprile 2009, il presidente Schifani mi rispondeva dando assicurazione circa la positiva evasione della proposta. A distanza di tanto tempo, e nulla essendosi ancora prodotto in tal senso, ho scritto nuovamente nei giorni scorsi al presidente Schifani per un sommesso sollecito, considerata la modesta entità prevedibile della spesa necessaria allo scopo e, viceversa, la doverosità - non solo formale del ricordo di un degnissimo uomo politico. Vorrei ora, portando le colleghe e i colleghi a conoscenza di questa mia iniziativa, chiedere l'appoggio di tutti perché in breve tempo si possa inaugurare l'opera.

del Paese, che seppe trovare, nella calda estate del 1982, una coralità di sentimenti e di orgoglio per un'Italia che si affermava agli occhi del mondo. Ieri mattina, si è spento a Milano, nella sua abitazione, Enzo Bearzot, commissario tecnico della nazionale italiana campione del mondo in Spagna Friulano di origine, come me e i senatori Pegorer, Saro, Lenna e Pittoni, è passato alla storia per la guida saggia, illuminata e vincente della nazionale azzurra dal 1975 al 1986. È un onore ricordarlo in quest'Aula, non solo come uomo di sport e figura carismatica del movimento calcistico, che ha dato a tanti la più grande gioia calcistica giovanile, ma soprattutto per il tratto umano, popolare, per la serietà dei suoi comportamenti, per la compostezza e la pacatezza, per il suo sapersi scostare dalle urla e dagli schiamazzi che troppo sovente caratterizzano in negativo il mondo del calcio e non solo quello. Le sue doti, che qui ho ricordato, Presidente, vorrei fossero esempio per il Paese e soprattutto per quanti lo rappresentano in tutte le sedi.

Prego,

Signor Presidente, desidero sostenere la proposta del collega Molinari di aggiungere il ritratto del senatore Giovanni Spagnolli a quelli degli altri Presidenti A dire il vero, non mi ero accorto di questa carenza nella galleria che è qui in Senato, ma con grande convinzione e affetto, anche conoscendone la famiglia, desidero unirmi a questa giusta rivendicazione, tanto più che Giovanni Spagnolli è stato l'unico trentino ad aver rivestito questa alta carica dello Stato, oltre a quella di Ministro della marina Inoltre, nel suo nome, la famiglia ha creato una fondazione, grazie alla quale si stanno realizzando grandi opere di carità in Africa. È una ragione di più per ricordarlo accanto agli altri Presidenti. **Sulla

Da avant'ieri, il Consiglio regionale della Sardegna è bloccato nella sua sessione di bilancio perché il Governo, per il secondo anno consecutivo, non comunica i dati formalmente consolidati con i lavori delle Commissioni paritetiche per la redazione delle norme di attuazione dello Statuto, che il Governo stesso ha inopinatamente richiesto, per la prima volta in sessant'anni. Si tratta dei dati che servono a a determinare il contributo dello Stato al funzionamento della Regione, cioè l'applicazione del nuovo regime delle entrate, che con una legge dello Stato, votata da questo Parlamento nel dicembre 2006, regola i rapporti tra lo Stato e la Regione Sardegna. È il secondo anno che questo avviene. Il presidente della Regione ha annunciato che sosterrà, con il parere favorevole di quella Giunta, una posizione che è una novità radicale, cioè la promozione di un conflitto di attribuzioni contro lo Stato italiano, contro il Governo, per questa radicale mancanza di lealtà e collaborazione. Per quanto riguarda i nostri lavori, segnalo che da settembre siamo in attesa, in Commissione finanze, che il Governo, come da impegno preso a novembre dal sottosegretario Giorgetti, venga per riferire formalmente la sua posizione. Signor Presidente, la prego di chiedere al presidente Schifani di aggiungersi alla richiesta già formalmente inoltrata da tutto l'Ufficio di Presidenza della Commissione finanze, ma rimasta inascoltata sino ad oggi, a circa

a proposito di quanto annunciato un momento fa dal senatore Gramazio, voglio sottolineare che tra le cause di questi drammatici crolli vi è la

manufatti assolutamente inadeguati, sia nel settore dell'edilizia scolastica che nel settore

Signor Presidente, voglio parlare di due fatti gravissimi che riguardano un colosso, l'ENI. Il primo fatto riguarda una perizia depositata nell'inchiesta per corruzione internazionale dai pubblici ministeri Fabio De Pasquale e Sergio Spadaro, secondo la quale l'ENI avrebbe pagato 187 milioni di dollari tra il 1994 e il 2004 per corrompere i politici nel Delta del Niger. Voglio ricordare che è una zona ricca di petrolio e che lì è stato impiccato Ken Saro-Wiwa, che difendeva il popolo degli Ogoni, che vive nel Delta.

Sono un senatore che desidera capire. Siccome ieri più volte il presidente Schifani nel suo intervento ha detto che i senatori ieri avevano difficoltà a capire, allora oggi voglio esercitarmi nel

tanto sbandierate da questa maggioranza. Ieri si è svolta una singolare riunione presso la sede della Provincia di Milano a cui hanno partecipato alcuni Comuni; segnatamente parlerò di un Comune della provincia di Milano e di quattro della provincia di Monza e Brianza.

Comuni interessati alla compartecipazione del 10 per cento, che sfiora i 50 milioni di euro (non stiamo parlando di noccioline), sono: il Comune di Carugate in provincia di Milano,